Onorevoli colleghi, come a tutti noto, nella giornata di ieri, a seguito di un tragico incidente stradale verificatosi sulla via Aurelia, nei pressi di Capalbio, è mancato il collega, senatore Altero Matteoli. La sua improvvisa scomparsa lascia sgomenti i familiari, gli amici e quella comunità politica e istituzionale di cui egli ha fatto parte per molti anni. Esponente di spicco della destra italiana, Altero Matteoli nasce a Cecina, in Provincia di Livorno, l'8 settembre del 1940. Egli inizia la propria carriera di dirigente politico del Movimento Sociale Italiano, di cui è segretario regionale in Toscana, nelle cui fila viene eletto a più riprese consigliere comunale e poi provinciale di Livorno. Dal 1983 è ininterrottamente parlamentare, prima alla Camera dei deputati e, successivamente, dal 2006, al Senato. Nel corso del suo mandato egli ricopre numerosi incarichi istituzionali: Ministro dell'ambiente nel primo, secondo e terzo Governo Berlusconi, nella XV legislatura diviene Presidente dei senatori di Alleanza Nazionale. Torna a ricoprire incarichi di Governo nel quarto Esecutivo Berlusconi, questa volta come titolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Dal 2006 al 2011 è altresì sindaco del Comune di Orbetello. Nel 2013 viene eletto Presidente della Commissione lavori pubblici e comunicazioni del Senato, carica alla quale è riconfermato il 21 gennaio 2016. Con Altero Matteoli scompare un parlamentare di indiscussa competenza e di grande esperienza, oltre che una persona dal tratto umano garbato e gentile. Viene inoltre a mancare un uomo politico che, pure orgoglioso della propria appartenenza culturale, è sempre stato in grado (come confermato anche dagli avversari più distanti), di unire alla rivendicazione delle proprie posizioni l'ascolto ed il rispetto di quelle altrui, insieme all'indubbia capacità di ricercare punti di equilibrio e di mediazione. Le considerazioni che immagino i Gruppi faranno saranno svolte nei prossimi giorni, in una commemorazione che sarà fatta alla presenza del famigliari. È probabile che le esequie di Altero Matteoli si celebreranno a Roma

Signor Presidente, credo che le riforme del Regolamento non si facciano solo scrivendo, ma anche nei comportamenti e pertanto, essendo previsto dal nostro Regolamento che la relazione debba essere consegnata e depositata cinque giorni prima (ma l'ho fatto un mese fa), credo che la prima regola debba essere che se c'è una relazione scritta a quella ci si debba riferire. Non intendo quindi aggiungere null'altro se non quello che dirò domani in sede di replica.

che cosa succederà se dovesse passare questa modifica del Regolamento, grazie anche al contributo che abbiamo dato: una svolta a nostro avviso epocale, avviso epocale, che prevede che finalmente le leggi di iniziativa popolare non saranno più insabbiate, non saranno più abbandonate nei cassetti stantii del Senato, com'è successo per la legge Parlamento pulito, com'è successo per la legge sull'acqua pubblica, leggi che sono state letteralmente abbandonate nelle Commissioni e mai discusse. Questa riforma del Regolamento prevede che tutte le leggi di iniziativa popolare, entro tre mesi, debbano essere portate in Assemblea, il loro lavoro deve essere concluso e portato ad un voto

Questa è una riforma a nostro avviso epocale. È una delle questioni sulle quali ci siamo battuti fin dal 2007, fin da quando abbiamo cominciato questa battaglia. Noi siamo nati con quel V-Day, con le leggi di iniziativa popolare per avere un Parlamento privo di condannati. Ecco, quel Parlamento privo di condannati era previsto nel testo di legge di iniziativa popolare: venne Beppe Grillo a portare il testo qui, a suo tempo. Sono passate due legislature - due legislature! - e la Commissione ha svolto lavori infiniti, audizioni Se questa riforma del Regolamento passerà, questa sarà la prima rivoluzione. Ma ce ne saranno tante altre, perché tante altre siamo riusciti, anche con il nostro contributo, a introdurre. La norma antitrasformismo: basta con i cambiacasacche. Avremmo voluto qualcosa di più forte, avremmo voluto che chi cambi il Gruppo parlamentare perda gli emolumenti che vanno al Gruppo. Quello era il nostro obiettivo, per evitare che si facesse un mercimonio del trasferimento di senatori da un Gruppo all'altro; che lo si facesse strumentalmente per ottenere un incremento economico delle dotazioni oppure oppure che ogni parlamentare, cambiando Gruppo, portasse con sé quella dote, che qui al Senato è di circa 60.000 euro, nelle spese del Gruppo. Purtroppo, non siamo arrivati a quel punto, siamo arrivati a un punto di caduta: almeno, abbiamo ottenuto che chi cambia casacca perda la poltrona degli incarichi avuti, come Presidente, Vice Presidente o Segretario delle Commissioni oppure Vice Presidente e Segretario del Senato. Cosa sarebbe successo se in questa legislatura avessimo avuto questo Regolamento? Regolamento? Forse la Presidenza del Senato sarebbe cambiata radicalmente man mano che passavano i mesi, considerato che abbiamo avuto la legislatura col più alto numero di cambio di casacche. Questa norma antitrasformismo consentirà di evitare che qualcuno faccia questi cambi nella prospettiva di avere premi con Presidenze, Vice Presidenze o altro. Queste sono due delle norme di buon senso. Gli altri colleghi, poi, racconteranno anche le altre: l'introduzione del voto elettronico, ad esempio, che, ovviamente, è prodromica all'introduzione anche dell'impronta digitale per evitare il fenomeno la possibilità di allattare (questo è uno degli emendamenti che sono stati proposti e che ci auguriamo qualcuno voglia accogliere): in questa legislatura ben due senatrici hanno avuto un bambino e hanno avuto la necessità di allattare e si è dovuta allestire una apposita sala sala per farlo, ma cosa c'è di più naturale del portare il proprio bambino in Aula? Cosa che, tra l'altro, già avviene al Parlamento europeo.

di audizione non siano pubblici: ecco, sopprimendo quel comma del Regolamento, i lavori possono diventare pubblici. Ovviamente, ciò non è automatico e la pubblicità dei lavori presuppone che vi siano poi altri interventi, ma questi potranno essere realizzati direttamente con delibera del Consiglio di Presidenza.

una questione che è stata sempre disattesa da questo Senato: quante volte abbiamo provato a introdurre dei disegni di legge in quota minoranza, che sono stati poi ignorati!

Signor Presidente, è che l'introduzione con i fatti che ha appena narrato sul collega Matteoli e l'improvviso intervento che mi è stato richiesto non

Quante volte in questo Senato abbiamo votato la dichiarazione d'urgenza di provvedimenti proposti dalla opposizione? Ovviamente, la maggioranza ha sempre lo strumento della Conferenza dei Capigruppo, in cui arriva il Capogruppo di turno il quale, con i numeri che porta alle sue spalle, decide la calendarizzazione a data certa dei provvedimenti. Le opposizioni che strumenti hanno? La dichiarazione d'urgenza, cioè chiedere che altri colleghi sostengano quell'urgenza e ogni volta anche quella viene disattesa. Ebbene, con questa modifica del Regolamento

un lavoro congiunto. È iniziato tutto dopo la bocciatura del *referendum* costituzionale, perché durante quella battaglia referendaria avevamo sostenuto più più volte che se si voleva rendere efficiente (non parlo di velocità, ma di efficienza) l'attività del Parlamento si poteva fare con delle piccole modifiche regolamentari.

gruppo limitato di persone può riuscire a elaborare un testo che sia il più possibile corretto e aderente al dettato costituzionale. Comunque siamo riusciti a introdurre un deterrente, per evitare che questo diventi uno strumento in mano alla maggioranza per fare molte più leggi: oggi infatti questo Paese non ha bisogno di più leggi, ma di meno leggi e di leggi migliori per far leggi migliori forse la Commissione è il luogo migliore. Abbiamo però introdotto dei deterrenti per impedire che questo diventi uno strumento abusato dalla maggioranza e cioè in qualunque momento, fino al voto finale, se un dato numero di senatori (un decimo per l'Assemblea o un quinto per la Commissione) si oppone alla prosecuzione dei lavori in quella modalità straordinaria si torna alla modalità ordinaria, con tutto il dibattito che ne consegue. Crediamo che questa questa modifica regolamentare sia un passo avanti. Non è il Regolamento che avremmo scritto noi: se lo avessimo scritto noi saremmo stati forse molto più duri e avremmo osato di più. È comunque un grande passo in avanti che forse segnerà una modifica dei lavori parlamentari

Prima di tutto, signor Presidente, vorrei rivolgere un ringraziamento al senatore Calderoli, al Comitato ristretto e a tutti i componenti della Giunta per il Regolamento per il lavoro svolto, per queste modifiche, sia pure parziali, del Regolamento, che sono tutte tese a cercare il massimo del consenso possibile in quest'Assemblea, cui talune disposizioni sono inevitabilmente frutto di una mediazione. Una mediazione che, se vista solo con riferimento alla singola disposizione, può generare generare qualche doglianza, qualche critica; ma se vista nel complesso, evidentemente si scolora rispetto all'obiettivo che tutti quanti noi abbiamo cercato di raggiungere. Sostanzialmente, queste modifiche del Regolamento tendono a una velocizzazione dei lavori parlamentari, in particolare dei lavori dell'Assemblea, il che, devo dire la verità, pone un primo un primo quesito, e cioè se questa velocizzazione fosse così necessaria a fronte di altre disposizioni, che prevedono invece una diminuzione del carico del lavoro

Una valutazione di massima positiva rispetto alle modifiche che vengono proposte mi consente di concentrare la mia attenzione solo in riferimento a talune disposizioni che, dal mio personale punto di vista, destano non poche perplessità. La prima la troviamo all'articolo 13, dove si dice che i Vice Presidenti e i Segretari che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Intanto, come giustamente segnalava la presidente Lanzillotta, le funzioni dei Vice Presidenti e le modalità di elezione degli stessi sono del tutto diverse da quelle che riguardano i Segretari. Mi chiedo, poi, cosa voglia dire che entrano a fare parte di un Gruppo parlamentare diverso. In altri termini, mi chiedo se la forma debba prevalere sulla sostanza, perché è chiaro che i Vice Presidenti e i Segretari possono votare continuamente in dissenso dal proprio Gruppo di appartenenza. Questo, che è un fatto importante e che evidenzia una lontananza del soggetto rispetto al Gruppo, non avrebbe valore rispetto a quanto prescritto dall'articolo 13. poi, il fatto che non so quanto questa disposizione in punto di sostanza possa essere sintonica con l'assenza di vincolo di mandato. È una disposizione complicata, questa, che trova un temperamento in un emendamento del relatore, il quale dice che la disposizione non si applica nel caso in cui il Vice Presidente o il Segretario entra entra a far parte di un Gruppo diverso non per una manifestazione di propria volontà ma per una manifestazione di volontà del Gruppo di appartenenza, che sostanzialmente lo espelle e lo allontana. Sul punto però vorrei fare una piccola evidenziazione. Il senatore Zanda, nel corso della discussione in Giunta per il Regolamento, ha difeso questa disposizione affermando che comunque i Vice Presidenti fanno parte dell'equilibrio maggioranza‑opposizione, così a mio avviso affermando una realtà che sicuramente è sintonica alla prassi ma non rispetto all'intero impianto istituzionale.

nel caso in cui dovessero manifestare la volontà di modificare Gruppo, perché questa disposizione non si debba applicare anche al Presidente del Senato. Può accadere, infatti, che il Presidente del Senato, eletto da una maggioranza,

Analogamente, c'è un'altra disposizione - che comprendo bene atteso il trasformismo che spesso connota la vita politica - che sostanzialmente impedisce la formazione di nuovi Gruppi parlamentari, salvo

i quali, si badi bene, devono prima di tutto rispondere ai loro elettori, che attraverso il loro voto hanno convalidato la loro elezione e, principalmente, hanno confermato la bontà del programma elettorale sottoposto al proprio vaglio. Credo che tale disposizione non sia corretta, nel senso e nei termini che poc'anzi ho rappresentato. Se un gruppo politico, ed evidentemente il Gruppo parlamentare di riferimento dovesse, per ragioni tutte interne al partito o al Gruppo, modificare seriamente la linea politica, davvero voi ritenete che legittima una norma che impedisca agli altri parlamentari di poter costituire un Gruppo autonomo che - si badi bene - trovi la sua ragione nella politica e non nel trasformismo della politica, della politica, ma nel rispetto del patto elettorale avuto con gli elettori e non dunque, come volgarmente si può dire, nella ricerca di posti e di *benefit*? Noi non possiamo legiferare la fisiologia, ancorandoci alla patologia che la prassi degli ultimi tempi ci ha rappresentato. Possiamo legiferare per contenere la patologia, ma non possiamo nel modo più assoluto comprimere i valori e gli ideali che ciascun senatore intende rappresentare.

Calderoli che il Presidente della Giunta per le elezioni debba essere un componente dell'opposizione,

mai quel Presidente dovesse entrare a far parte della maggioranza, decadrebbe. Ma cosa vuol dire entrare a far parte della maggioranza? Vuol dire dichiarare espressamente un cambio del Gruppo? Vuol dire votare sintonicamente tutti i momenti insieme con la maggioranza? Vuol dire, ad esempio, votare la fiducia al Governo? Io credo, trattandosi della Giunta per le elezioni (ma il ragionamento si potrebbe fare per qualsiasi altro organismo di garanzia), che questa norma debba essere più specifica e precisa, perché secondo me non si può consentire che un organo di garanzia venga presieduto da un camuffato membro della maggioranza. Se si devono fare modifiche al Regolamento, esse devono essere serie, approfondite e tali da funzionare

Intanto questo pone un primo problema, e cioè che i Gruppi dovrebbero essere particolarmente attenti nella composizione delle Commissioni perché, essendo diverse le sensibilità che vi sono all'interno di ogni Gruppo, ove queste sensibilità fossero rappresentate in maniera squilibrata e sproporzionata all'interno della Commissione,

ma guardate che dare la possibilità di tornare alla sede normale, cioè di superare sia la sede redigente che la sede deliberante, significa sostanzialmente non modificare nulla, e cioè rendere le cose così come esse attualmente sono; quando invece sarebbe stato preferibile, come oggi è, che la sede deliberante fosse il frutto di un accordo delle forze politiche. Perché io sono certo che, nel momento in cui non si dovessero registrare dei punti di convergenza in Commissione, per qualsiasi disegno di legge con riferimento al quale questo punto di convergenza non si dovesse verificare, partirà la richiesta di tornare al lavoro normale in Assemblea. Ancora, vi è una disposizione che riguarda sostanzialmente l'illustrazione e la presentazione degli emendamenti: è una modifica all'articolo 100.

i lavori; ma se per ipotesi all'interno di tutti quegli emendamenti vi fosse un emendamento presentato da uno dei senatori del Gruppo in totale dissenso con il Gruppo stesso, quel senatore non avrebbe all'attualità della modifica alcuna possibilità di illustrare l'emendamento. So perfettamente che il senatore Calderoli ha preparato una riformulazione di un emendamento presentato dal senatore Malan, che a mio avviso era molto più rispettoso dei diritti dei senatori e della loro prerogativa di esercitare la propria funzione senza vincolo di mandato. Però, come ho già detto al senatore Calderoli in sede di Giunta per il Regolamento, la sua riformulazione non è soddisfacente fino in fondo: fondo: se è vero che consente al presentatore di un emendamento in dissenso la possibilità di intervenire, è altresì vero che nel caso in cui gli emendamenti in dissenso fossero più di uno, e più di uno fossero i presentatori, solo uno di questi presentatori avrebbe la possibilità di parlare, e non necessariamente quel presentatore in dissenso potrebbe avere sugli altri emendamenti una visione sintonica a quella degli altri presentatori.

diamo un primato di autorità - non di autorevolezza - ai partiti. che questo non sia assolutamente un fatto positivo. Né si può dire che il presentatore di un emendamento in dissenso ha comunque la possibilità di parlare in dichiarazione di voto, evidentemente in difformità rispetto alla dichiarazione del Gruppo. Gruppo. Affermare una cosa di questo genere significherebbe sostanzialmente dire che la fase dell'illustrazione degli emendamenti non serve assolutamente a nulla, quando tutti noi sappiamo che quella fase dell'illustrazione degli emendamenti, specie se non abusata, è il momento in cui si può spiegare ai senatori e all'Assemblea le ragioni di un emendamento e, se del caso, come spesso è accaduto in quest'Aula, convincere i senatori di un'altra parte politica a votare quell'emendamento. Quante volte è accaduto? Tutto questo viene compresso in ossequio al *totem* della velocità

C'è un emendamento secondo cui i lavori del Senato dovrebbero prevedere anche la possibilità dell'ingresso dei lattanti per l'allattamento. Intanto, correggerei quell'emendamento perché mi pare che la maternità e la paternità siano equiparate e, se è vero che il papà non può fisiologicamente allattare, è altresì vero che lo può fare in tutti i casi di allattamento artificiale. Non potete affermare una cosa di questo genere senza alcuni correttivi. Davvero ritenete che l'allattamento

altri? Conseguentemente, l'allattamento in Aula non è esattamente la strada migliore per venire incontro alle esigenze della maternità, ben potendosi sospendere il lavoro per quindici o venti minuti e consentire alla mamma di allattare il figlio nel modo che ella ritiene più opportuno. Scusate, ma quando la mamma allatta in Aula il circuito radiotelevisivo è in funzione? I fotografi dalle tribune svolgono Tutto questo lo ritenete rispettoso della donna, specialmente di quella donna che volendo, per ipotesi, allattare in separata sede

di sentirmi dire a ogni piè sospinto «ce lo chiede l'Europa». Ma, insomma, vi rendete conto che l'Europa è un qualcosa di inafferrabile ormai, con oltre venti Paesi che ne fanno parte, molti dei quali con tradizioni e storie completamente diverse dalle nostre? nostre? Una cosa è andare a regolamentare i capisaldi di determinati settori e una cosa ben diversa è incidere sul costume di un popolo. «Ce lo chiede l'Europa»: l'Europa non l'ha fatto. europeo nel proprio regolamento assembleare non ha una disposizione di questo genere. Se del caso, è una norma che può essere varata dal Consiglio di Presidenza nei

quali siano i casi eccezionali e se davvero, di fronte a una eccezionalità del caso, la necessità dell'allattamento

Davvero anche in questo caso, secondo voi, la velocità deve fare strame delle sensibilità strame delle sensibilità che accompagnano la donna in uno dei momenti più belli e più delicati della sua vita?

l'occasione anche per ringraziare il Presidente Grasso, che finalmente si è ricordato che presiede la Giunta per il Regolamento.

fortunatamente è entrato in politica e si è svegliato pure lui. Ho presentato tre emendamenti sulla proposta

le controversie si concludono poi nella legislatura qualcuno deve pagare. Poi ne ho presentati altri due, uno sul rendiconto analitico della spesa dei senatori - visto che anche in Consiglio di Presidenza ho portato questo argomento, ma si fanno orecchie da mercante - e l'altro per i collaboratori dei parlamentari, che, come abbiamo visto, spesso vengono assunti, ma non vengono pagati e anche di questo si discute solo a fine legislatura. Avevamo cinque anni per risolvere alcune questioni, non lo si è voluto fare e mi auguro che il nuovo Regolamento in qualche modo possa modificare l'andamento

di alto idealismo. Invito però entrambi i senatori, rappresentanti del Movimento 5 Stelle, ad avere un attimo di pudore. Va benissimo benissimo incidere sul Regolamento del Senato, perché sono i Regolamenti che hanno fatto evolvere la democrazia, da Atene al periodo della Magna Charta, a tutte le modifiche del Regolamento e dei Gruppi parlamentari che ci sono state dall'inizio

È importante incidere sui Regolamenti, perché essi permettono di legiferare bene, di dare una rappresentanza popolare e di far sì che i parlamentari siano effettivamente voce della Nazione e del popolo

Il Movimento 5 Stelle, che tanto fa esaltazione della democrazia diretta e poi non la applica neanche all'interno del Gruppo, dovrebbe allora fare un *j'accuse* perché non ha rispettato neanche il neanche il regolamento del suo statuto depositato in Senato. Infatti, alla faccia della democrazia e del rispetto degli alti ideali, in questo Senato sono state espulse dal Gruppo ben 19 persone - 19 senatori - e

le *chat* o le conversazioni e fare dossieraggio. È molto difficile intervenire in quest'Aula dove c'è l'autodichia;

che non vengono mai citati quando, ad esempio, si fa tanto populismo guardando le bricioline dei costi del parlamentare o quando si fanno le rendicontazioni finte, oppure talmente

precisi allo 0,01. Voglio dire che per essere democratici bisogna essere anzi tutto trasparenti e coerenti e far sì che un regolamento, se ci deve essere, sia anche, di conseguenza, rispettato. Dobbiamo anche dire che si è fatto sempre populismo sulle trasmigrazioni e a tale proposito ci sono quelli che sono usciti volontariamente e ci sono quelli che invece sono stati espulsi, che è una cosa molto diversa. Io personalmente sono stata espulsa, diciamolo chiaramente. All'interno del Movimento 5 Stelle avrei rotto le scatole continuamente e fino alla fine perché le cose che avevamo promesso non le abbiamo poi applicate: lo dobbiamo dire che le cose sono andate un po' diversamente, che sono stati presi in giro quei famosi nove milioni di elettori. Lo Lo dobbiamo dire che, in realtà, non siamo stati una riduzione dei costi per la politica, perché abbiamo speso tantissimo e di quei soldi si è fatto anche un uso discutibile e privato. Mi riferisco all'ufficio di comunicazione esterno che decide, non è soltanto un mero ufficio di comunicazione ma dà una linea politica, una direzione politica; quindi il popolo viene sostituito da un gruppo ristretto in una stanza

tempi doveva essere tutt'altro. Quindi, da un lato, bisogna rispettare la linea del Gruppo, come è giusto che sia, perché vi è un programma con cui uno si presenta; dall'altro, ogni parlamentare è parlamentare della Nazione. C'è anche da dire che, purtroppo, ora le cose sono molto più confuse, perché non abbiamo quegli schieramenti, quel bipolarismo classico: conservatori-rivoluzionari, destra-sinistra; tutto è più confuso

tratta di una restituzione: rinunciare a certe cose, per pagare i funzionari, il personale, le segreterie, con la propria quota di 6.000 euro, che è più che sufficiente, credo, per contribuire a un Gruppo.

a espellere il parlamentare, senza un motivo valido, non rispettando le regole che lo stesso Gruppo parlamentare si è dato e ha depositato in Senato, in quel caso deve essere il Gruppo a pagare; pagherà al parlamentare la stessa cifra, ovverosia una quota proporzionale ai mesi di permanenza del parlamentare nel Gruppo. Dopodiché, il parlamentare porterà quella quota nel Gruppo cui accederà.

a rispettare le regole e a non fare le famose trasmigrazioni che avvengono così spesso (i famosi cambi di casacca). è il Gruppo parlamentare a buttare fuori dei parlamentari, per quante volte lo può fare, in infrazione al regolamento del Gruppo? Secondo me non un numero infinito di volte. Pertanto ho proposto che, oltre i tre parlamentari espulsi al di fuori delle regole (quindi non rispettando le regole che il Gruppo stesso si è dato e che ha depositato in Senato), il Gruppo debba considerarsi automaticamente sciolto e i parlamentari debbano debbano confluire nel Gruppo Misto. Il Gruppo Misto, a mio avviso, non deve essere fatto di tante componenti; ognuno, se ha il suo pensiero particolare, se lo tiene, ma il Gruppo Misto deve essere misto, neutro, senza componenti.

più uguaglianza e più opportunità per tutti, che siano tutti un po' più liberi e tutti un po' più uguali. Concludo, signor Presidente, citando Max Weber, il quale sosteneva che ci sono due modi di fare il politico: si può vivere per la politica oppure si può vivere della politica. Ecco, spero che il nostro Regolamento venga modificato in modo tale che nessuno viva più della politica, a scapito di chi, eletto, vive per la politica. PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'argomento in discussione oggi è sicuramente uno dei più importanti e delicati affrontati in questa legislatura. Lo è, prima di tutto, per la peculiarità dell'organo legislativo, ma - ancor di più - se si considera il mancato voto favorevole al *referendum* costituzionale del 2016. Infatti, è passato esattamente un anno dal famoso 4 dicembre e finalmente ci si è resi conto che intervenire sulla tempestività del procedimento legislativo, sull'armonizzazione e sul riordino di talune procedure parlamentari è non solo necessario (lo è sempre stato e - azzardo a dire - lo sarebbe stato anche in caso di vittoria dei sì), ma - ora - addirittura indispensabile. Pertanto, giungo a dire: finalmente. Finalmente la revisione del Regolamento. Ben venga, quindi, il confronto su questo tema. Al contempo, è giusto anche dare una serena valutazione sul come si sono svolti i lavori parlamentari nell'attuale legislatura in relazione all'applicazione dell'attuale Regolamento interno. Diciamo che il Regolamento ha mostrato tutti i suoi limiti e non si sono potute evitare lungaggini varie, distorsioni regolamentari, persino abusi interpretativi anche a fini ostruzionistici, o eccessiva rigidità delle disposizioni in esso contenute. Era dunque inevitabile e attuale un processo di revisione. Regolamento del Senato proposta dal presidente Grasso rappresenta, quindi, un passaggio importante che - mi auguro - terrà conto del parere di tutti i Gruppi parlamentari e anche dei singoli senatori. Da parte mia, ho voluto dare il mio contributo, integrando il testo proposto dalla Giunta per il Regolamento con alcune modifiche, quali ad esempio la previsione di un codice di condotta dei senatori, già in parte introdotto alla Camera dei deputati. Tale richiesta proviene sia dal Consiglio d'Europa, che dall'OSCE. Ricordo, infatti, la Dichiarazione di Bruxelles dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, la quale, già nel 2006, all'articolo 12 della risoluzione sui limiti all'immunità parlamentare al fine di rafforzare la buona *governance*, l'integrità pubblica e lo Stato di diritto nella regione dell'OSCE «incoraggia i Parlamenti degli Stati partecipanti dell'OSCE a: definire e pubblicare rigorose norme di etica e di condotta ufficiale dei parlamentari e del relativo personale; personale; creare meccanismi efficienti di pubblicità delle informazioni finanziarie e dei potenziali conflitti di interesse dei parlamentari e del relativo personale; creare un ufficio di *standard* pubblici al quale si possano presentare reclami per le violazioni degli *standard* da parte dei parlamentari e del relativo personale; creare procedure efficaci e tempestive per indagare su tali reclami e per prendere provvedimenti disciplinari nei confronti dei parlamentari e del relativo personale qualora essi siano accolti». Questo riferimento all'OSCE va in parallelo alla recente valutazione fatta dal GRECO (Gruppo di Stati contro la corruzione), organo del Consiglio d'Europa, pubblicata lo scorso 19 gennaio, gennaio, sul sistema italiano nella prevenzione della corruzione tra i membri del Parlamento, con specifico riferimento al Senato italiano e alla necessità da parte di quest'ultimo di adottare un codice di condotta, sulla scia di quanto già fatto alla Camera dei Deputati. Ricordiamoci, infatti, che la Camera ha un codice di condotta, mentre

alle sue disposizioni; effettive disposizioni sanzionatorie». Queste misure sono raccomandate anche per il Senato. Ritengo pertanto imprescindibile prevedere norme che prevengano e rimuovano situazioni di conflitto di interessi, con adeguate sanzioni, anche di carattere pecuniario, da applicare a chi non rispetta non rispetta tali disposizioni. In particolare, ogni senatore, nell'esercizio del proprio mandato parlamentare, dovrà essere guidato dai principi di onestà, integrità, trasparenza, responsabilità, diligenza ed esemplarità, a tutela del buon nome dell'istituzione che rappresenta. [**Presidenza della vice presidente anche l'inserimento di criteri comportamentali di serietà e rispetto dell'altro, nonché principi di sobrietà e trasparenza. A mio modesto parere devono essere valori e condotte comuni a tutti i membri del Parlamento (ricordo anche l'articolo 54 della nostra Costituzione, riferito alle persone che hanno cariche pubbliche e che devono adempiere al loro mandato con disciplina e onore), non solo *slogan* propagandistici di un partito o movimento politico. A proposito di definizioni, sono intervenuto nello specifico all'articolo 14, comma 4 della proposta di modifica, perché credo sia inutile e fuorviante inserire un esplicito riferimento ad un concetto come quello di movimento politico. Ritengo che prendendo come fonte principale del Regolamento la nostra Costituzione, questa cita solo i partiti politici quali attori della politica italiana e non usa altri termini. Inoltre, se pur volessimo considerare quanto previsto nella legge elettorale in vigore, ovvero la n. 165 del 2017 (il cosiddetto Rosatellum-*bis*) in questa si fa riferimento, all'articolo 4, quando si parla di elezioni trasparenti, a «partito, movimento e gruppo movimento e gruppo politico organizzato che ha presentato le liste», aggiungendo anche la dizione di gruppo politico, non prevista dalla nostra modifica del Regolamento che si limita a partiti e movimenti politici. Stiamo escludendo quindi i Gruppi politici. politici. Per semplicità, dunque, ma anche per evitare differenti interpretazioni sull'assenza dei Gruppi politici previsti nella legge ma non nel Regolamento utilizzerei un unico termine per indicare chi ha diritto di avere la rappresentanza parlamentare organizzata in Gruppi parlamentari, ovvero i partiti,

Inoltre, non potevo non fare riferimento, anche in questa occasione, alla necessità di adottare un quadro disciplinante per la rappresentanza di interessi, al fine di rendere chiare e trasparenti le fasi del processo decisionale, nell'interesse dei cittadini. Disciplinare, quindi, i rapporti fra lobbisti e decisori pubblici rappresenta un passo fondamentale per lo sviluppo socio-economico del nostro Paese. Su questo, come noto, la Camera dei deputati, anche in quel caso, ha introdotto disposizioni per ora assenti al Senato. Questa è l'occasione buona per farlo,

e che andrebbe regolamentata. Infine, mi sono sentito in dovere - anche in virtù della mia esperienza personale - di introdurre un'eccezione che salvaguardasse la democraticità interna dei Gruppi. Infatti, il combinato disposto degli articoli 13 e 27 della proposta di modifica rischia di soffocare la pluralità di voci e punti di vista all'interno di un Gruppo parlamentare: essere espulsi da un Gruppo,

in generale vanno nella direzione giusta, ma ci sono delle gravi lacune e carenze che in questo mio intervento ho illustrato e che con i miei emendamenti potranno essere sanate. Mi riprometto, nel corso dell'illustrazione degli emendamenti, di

Signora Presidente, innanzitutto, vorrei criticare il fatto che si proceda a una modifica del Regolamento in una fase così a ridosso di una nuova legislatura. Oltretutto, una nuova legislatura che verrà avviata con una legge elettorale di cui nessuno può dire quali potranno essere

tra eletti e volontà degli elettori, tra rappresentanti e rappresentati. Quindi, mi permetto di fare questa critica perché agire su una imminente nuova legislatura,

in questo Senato. Ma vale sempre il detto: chi la fa l'aspetti. Quindi, prudenza vorrebbe che, nel momento in cui ci si accinge a cambiare le regole per qualcun'altro, ci si mettesse in una condizione ipercritica, ipercauta e anche

omogeneo, più regolare, anche più approfondito, un lavoro in cui può esservi un maggiore bilanciamento tra quei momenti di approfondimento che, inevitabilmente, avvengano nelle Commissioni e il momento della discussione plenaria dei provvedimenti.

quelli che il popolo si è abituato ormai a sentir definire come cambi di casacca. L'incoerenza, sicuramente, è un fatto grave, soprattutto in chi si prende la responsabilità di rappresentare altri. Ma vede, senatore Calderoli, l'incoerenza non è un comportamento che può essere impedito per legge, perché l'incoerenza è una devianza rispetto a un valore morale che dovrebbe essere, invece, la missione più importante, più lucida e più chiara per chi chiede di essere votato per poi venire qui a rappresentare delle idee e dei pensieri. Non è neanche legittimo confondere il concetto di dissenso con il concetto di cambio di gabbana, come spesso è stato definito un comportamento che forse non è stato possibile chiarire o è stato male riportato o, forse, è stato anche strumentalizzato. Infatti, senatore Calderoli,

che la Costituzione, con l'articolo 67, relativo alla libertà di mandato, intenda tutelare con grande fermezza il rapporto coerente, trasparente e veritiero che l'eletto deve avere nei confronti dei propri elettori, i quali sono ovviamente nella condizione di valutare solo un programma elettorale e su quello dare la loro fiducia.

di tutelare la propria posizione e di poter accedere agli atti per verificare la veridicità delle dichiarazioni dell'allora capogruppo Santangelo sulla conformità dei provvedimenti presi nei confronti di ben nove senatori senatori rispetto allo statuto e al regolamento che il Gruppo aveva depositato e che, a mio avviso, fanno parte integrante del *corpus* con cui si governa quest'Assemblea e con cui ciascun Gruppo si regola.

credo sia il segnale più grande di come oggi, nel momento in cui siamo di fronte a una riforma del Regolamento, dobbiamo prendere precauzioni ed essere attenti a non confondere il legittimo dissenso e la dialettica che legittimamente un rappresentante del popolo, che prima di tutto è un rappresentante del popolo, deve potersi vedere garantiti all'interno di questa Assemblea: non solo all'interno del proprio Gruppo, ma anche all'interno di quest'Assemblea e questo non viene tutelato nella modifica regolamentare.

fortemente gerarchica la relazione che all'interno dei Gruppi si instaura tra chi dirige il Gruppo

che sono stati spostati proprio in relazione a una non affidabilità che l'espressione della loro opinione poteva avere rispetto alla linea decisa dal partito, in una logica di numeri che è inaccettabile in quanto la logica dei numeri, che è nella disponibilità dell'elettorato, si consuma all'interno delle urne elettorali e nella scelta di singoli rappresentanti.

del sistema elettorale. Si tratta allora di una sublimazione di questo assetto gerarchico. Mi fa effetto vedere che, di fronte a questa sublimazione, si scateni l'entusiasmo del Gruppo «uno vale uno»; di quell'uno vale uno che doveva essere a suo tempo, ma come si cambia per opportunità! Questa logica gerarchica è ripercorsa con malizia in tutti i dettagli del legiferare. Viene ricondotta in sostanza a negoziati che vengono fatti in altra sede, a negoziati basati sulla forza, quando proprio il mio ex Gruppo si è ripetutamente, per cinque anni, lamentato della non volontà dei colleghi senatori

ci troviamo qui a discutere della riforma al Regolamento. Mi soffermerò esclusivamente su due punti che mi stanno particolarmente a cuore e che, se la riforma del Regolamento verrà approvata, così come sembra, potrebbero migliorare, anzi miglioreranno sicuramente l'andamento dei lavori a partire dalla prossima legislatura.

non molto bello a vedersi, che è il Regolamento del Senato, e vidi che all'articolo 115 c'era una disposizione che prevedeva la votazione elettronica. Cosa significa? Che ciascun senatore può votare premendo uno dei tre pulsanti che indicano se si astiene, se è contrario o favorevole. Per fare in modo che questo meccanismo venisse utilizzato un senatore si doveva alzare e chiedere ogni volta il voto elettronico. Così ho iniziato a fare, e i primi mesi l'ho fatto almeno centinaia di volte al giorno. Lascio immaginare le risa da parte di tutti quanti, perché non avrebbero immaginato il mio perseverare nella richiesta,

Grazie

Questa misura, all'interno del Comitato ristretto, che si è adoperato per cercare di fare una sintesi rispetto a tutte le proposte, non è stata accettata, ma le Commissioni possono decidere

gli italiani avevano bisogno in questo momento storico di una riforma del Regolamento del Senato? Forse sì, ma forse anche no. Probabilmente, se la stessa attenzione fosse stata posta su argomenti di gran lunga più importanti, come il reddito di cittadinanza o una seria legge anticorruzione, probabilmente il lavoro che noi tutti potevamo portare

Signora Presidente, io devo innanzitutto complimentarmi con la Giunta per il Regolamento, perché a una prima lettura delle modifiche mi sembrava di poterle condividere tutte. Ad una seconda lettura, invece, mi sono sorti alcuni dubbi. Devo dire, senatore Calderoli, che nel dibattito che c'è stato finora ho colto ulteriori spunti di riflessione che mi erano sfuggiti: ad esempio, ho apprezzato e apprezzo le modifiche relative ai tempi di discussione e di decisione; e apprezzo il collegamento dei Gruppi parlamentari con le liste.

senatori decidono di uscire dai rispettivi Gruppi per fare un nuovo Gruppo...

Dovremmo restare nei rispettivi Gruppi, ancorché facciamo un Gruppo a parte. Poi avremo Poi avremo sanzioni disciplinari dai Gruppi, ma ci comporteremo secondo la logica della condivisione di una determinata posizione.

una semplice limitazione individuale, ma una limitazione addirittura di dubbia costituzionalità sotto il profilo della rappresentanza di un Gruppo politico, quindi di un'espressione politica già esistente. Presidente Zanda, al Gruppo Articolo 1-MPD, di cui è entrato a fa parte anche il Presidente del Senato, neghiamo la legittimità perché non è collegato a una lista presentata alle elezioni? Ho qualche serio dubbio che possa essere accettata una soluzione di questo tipo.

la filosofia della nostra Costituzione. Senatore Calderoli - mi rivolgo a lei perché è relatore e non perché è responsabile di queste soluzioni

per illustrare tutti gli emendamenti. A parte l'impossibilità di illustrare in dieci minuti tutti gli emendamenti, consideriamo il caso in cui vi sia un mio emendamento in contrasto con il Gruppo.

Come oggi mi sono convinto delle osservazioni fatte dal senatore Palma, può darsi che quelle osservazioni convinceranno qualcun altro. Vi rendete conto che con questa forte limitazione delle possibilità dal singolo senatore

perché non ha avuto il consenso necessario da parte di ciascun Gruppo e di ciascun senatore.

ritengo che il procedimento legislativo non vada accelerato, perché stiamo producendo troppe leggi. Questo è lo stesso errore della riforma costituzionale, bocciata dal popolo italiano. Anche quella riforma si fondava sull'erronea convinzione il Parlamento producesse troppe leggi. No, il Parlamento produce troppe leggi sbagliate, al punto tale che anche l'ultimo documento del procuratore della Repubblica, a proposito delle intercettazioni, ha detto ai parlamentari: fermativi; non approvate più leggi. Non è una posizione isolata dei procuratori della Repubblica. Consultate gli operatori del diritto, dagli avvocati, ai notaio, ai magistrati. Dicono che stiamo producendo una marea di leggi,

una serie di norme su cui è difficile anche fare un minimo di riflessione. Pertanto, come si può pensare

Riducete i tempi, ma non eliminate la possibilità di intervento, non eliminate la possibilità di suggerire soluzioni diverse, perché soltanto da un confronto reale le leggi possono essere conformi

come risolvere il problema? Io credo che vada confermato il collegamento di ciascuno di noi con i Gruppi di elezione.

ad una opzione politica diversa, come se fosse un partito diverso, e lo è diventato. Come si fa a dire no perché non è ricollegato ad una lista di elezione? Questo è uno dei punti che bisogna correggere. Ho svolto due osservazioni: questa e quella relativa alla sede del procedimento legislativo, che va confermata in alcuni aspetti e corretta per altri. riuscire veramente a fare un discorso di funzionalità, perché questo testo, così com'è stato varato, non determinerà funzionalità sotto il profilo del procedimento legislativo. Invece, con quelle correzioni credo che potremmo rendere un servizio al Paese, prevedendo una nuova forma di partecipazione alla vita del Senato tale da garantire un

del confronto. Alla base di quel testo vi è un confronto tra le varie forze politiche al fine di individuare una soluzione; a meno che non si voglia fare come io ho ripetuto varie volte in Commissione, in Commissione, dove si adotta una tecnica che è completamente contraria a quella degli organi collegiali. La maggioranza vota, si può fare qualsiasi osservazione ma nessuno risponde.

Questo potrà avvenire anche in Aula e sarebbe una tragedia per la nostra Repubblica! Signora Presidente, colleghi, io credo che nell'analisi di questo documento di modifica del Regolamento, dovremmo porre attenzione a qual è il ruolo che vogliamo assegnare al Parlamento e al Senato nella fattispecie: se, come ho visto tantissime volte, esso deve essere semplicemente la cassa di risonanza del Governo e delle organizzazioni partitiche o se, invece, deve essere effettivamente un luogo di elaborazione e di decisione per ottenere una normativa non solo più velocemente ma anche qualitativamente più efficace. Se noi leggiamo la maggior parte delle leggi che sono state approvate negli ultimi anni, possiamo concordare, senza grandi problemi, sul fatto che esse sono scritte male, perché di difficile comprensione e necessitanti di un'interpretazione laboriosa, talvolta complicata anche per gli operatori del diritto. Sicuramente, quindi, serve una produzione normativa più chiara e più leggibile, migliore, non necessariamente più veloce. Questo non vuol dire che l'attività debba essere lenta e che quest'Assemblea debba diventare improduttiva.

la riduzione degli spazi di intervento nei processi da parte dei singoli membri di questa Assemblea. Questo, purtroppo, mi pare che sia lo spirito complessivo della modifica che ci accingiamo a votare. Io vengo da una storia molto complessa, così come alcuni colleghi che mi hanno preceduto, all'interno di un Gruppo parlamentare che pochissimo o nessuno spazio dava al dissenso. Se noi immaginassimo di annullare - così come quel Gruppo pensa di fare - il divieto di mandato imperativo e quindi statuire (dovrebbe essere fatto in Costituzione) che il parlamentare deve adeguarsi a quanto disposto, al momento del mandato, dal partito, partito, questo tipo di modifica e questo tipo di percorso potrebbero avere un senso. Ma se noi riteniamo che ognuno di noi debba esprimere, in scienza e coscienza, la propria opinione e il proprio voto sui temi che gli vengono proposti, la cosa diventa più complessa. Vedete, ciò che la gente chiede, da quanto ho potuto capire in questi cinque anni, è che gli impegni che i partiti assumono nei confronti del proprio elettorato vengano rispettati. Il problema è che spesso i partiti non fanno così. Per i motivi più vari, può capitare che un partito che, ad esempio, aveva preso l'impegno di far valere

A questo punto, il parlamentare che intende attenersi agli impegni presi con l'elettorato (da cui effettivamente dovrebbe dipendere) al momento dell'elezione cosa dovrebbe fare? fare? Seguire il nuovo modo di pensare, le nuove decisioni del partito cui ha aderito, quindi seguirlo in questo allontanamento dal mandato del partito, o rispettare il mandato che aveva assunto con gli elettori all'inizio? Ritengo che debba fare questa seconda cosa. Ma a questo punto, perché penalizzare... penalizzare il gruppo di parlamentari che, attenendosi al mandato iniziale, chiede di continuare la propria attività sotto quel segno? Penso che sia utile una discussione e ascoltarci reciprocamente durante questa discussione generale, per ottenere un risultato ottimale per questa modifica del Regolamento, che può essere una buona occasione per migliorare il lavoro di questa Camera.

avere un approccio che coinvolge tutte le forze politiche nel fare piccole o grandi riforme delle nostre istituzioni. si può fare a condizione di avere un approccio pragmatico e cercare di fare delle regole che soddisfino meglio le esigenze delle istituzioni, in questo caso del Senato, e non fare la convenienza di parte. Credo che se in futuro si ritornerà - io spero di sì - di sì - a pensare a riforme della Costituzione, bisognerà lavorare con il metodo con cui si è lavorato su questa riforma del Regolamento e non con quello adottato nella parte precedente della legislatura per la riforma della Costituzione che, non a caso, è stata bocciata dagli italiani. Venendo al contenuto della riforma in esame, l'intendimento è quello di rendere i lavori più efficienti e rapidi

ma non si può impedire a nessuno di questi senatori di passare a un Gruppo della parte opposta. Pertanto, un senatore eletto a sinistra non avrà alcuna difficoltà a passare a un Gruppo di destra, il che - insomma - è un po' incongruo rispetto all'altra proibizione.

caso ipotetico, che spero resti tale, perché credo che la fisiologia dovrebbe essere che un movimento politico si presenti alle elezioni e che suoi rappresentanti, con qualche divergenza al loro interno, restino nel Gruppo e si esprimano nel corso delle votazioni. Ma quando questo non succede, però, vorrebbe dire che questo Gruppo Misto, dove ci sarebbero persone di destra, di sinistra, di centro, provenienti avrebbe diritto a esprimere una sola dichiarazione di voto in una serie importante di circostanze senza dare conto alcuno della varietà di rappresentanze che può avere e che, anzi, anche oggi stesso ha al

non si tratta soltanto di tutelare il dissenso, perché non c'è soltanto quello, ma ci sono anche i punti diversi che possono emergere negli emendamenti ad un solo articolo.

ordinariamente l'articolo è uno solo, perché se si riforma un articolo del codice penale, sarà uno solo l'articolo che lo esprime. Ci può quindi essere non soltanto dissenso, naturalmente anche questo,

non confidare troppo, nel cambiare le norme, nel fatto che poi ci sarà la discrezionalità della Presidenza, perché altrimenti manteniamo la discrezionalità e lasciamo stare le regole. Sappiamo che difficilmente un Presidente direbbe di no

e in dichiarazione di voto, magari in dissenso, ma anche senza il dissenso, perché le regole sono le stesse, quindi tutto quello che vediamo in Assemblea dovrebbe essere applicato in Commissione,

non per irrigidirle al punto da rendere necessario o addirittura indispensabile in certi casi derogare a queste regole. Io sarei per avere meno regole e nessuna deroga, piuttosto che più regole regole e tante deroghe. Detto questo, nel ringraziare i membri della Giunta per il Regolamento per il lavoro che hanno svolto in Commissione, anche in sede di esame degli emendamenti presentati per l'Assemblea, io conto che ci sia un ulteriore approfondimento e miglioramenti nell'ambito della discussione degli emendamenti che verranno esaminati domani.

io credo che la XVII legislatura, nata senza maggioranza parlamentare, almeno in questo ramo del Parlamento, verrà ricordata, quando il tempo della cronaca politica lascerà spazio alla piccola storia parlamentare, come una legislatura importante, non solo per i provvedimenti approvati o per il sostegno a Governi che hanno aiutato il Paese in un frangente difficile della propria storia, ma anche e soprattutto come una legislatura responsabile, che in numerose occasioni ha visto prevalere tra noi il senso e la necessità delle cose da fare, per il bene comune, al di là della normale dialettica tra le parti. parti. Lasciatemi dire che questo spirito di responsabilità traspare anche da questa riforma del Regolamento, che spero tutti insieme approveremo nella giornata di domani. Vorrei davvero riuscissimo tutti a far emergere fuori da qui, in quella che probabilmente è la nostra ultima settimana di lavoro parlamentare, un atto, non solo di responsabilità ma - mi si consentirà il termine - di affetto nei confronti delle istituzioni. Per questo è giusto ricordare l'impegno del Comitato ristretto, composto dai colleghi Bernini, Buccarella, Calderoli e Zanda per una ragione che quest'Assemblea consegna alle prossime legislature, privilegiando un atto che certamente non avrà per i nostri partiti alcun impatto elettoralistico e per il quale certamente nessun cittadino si fermerà per strada a ringraziarci, ma che vuole, a distanza di quarant'anni dalle riforme del 1971, aggiornare uno strumento decisivo per il buon funzionamento delle istituzioni parlamentari. Un nuovo Regolamento - lasciatemelo dire - che affonda le proprie radici nel lavoro svolto in legislature precedenti. Voglio qui riconoscere proprio alla proposta Zanda-Finocchiaro, presentata ormai qualche anno fa, il merito di essere stato il canovaccio sulla base del quale tutti ci siamo mossi in questi mesi. una riforma che credo faciliterà il confronto politico, all'interno di un sistema per la prima volta tripolare, anche se nella propria applicazione dovrà tener conto del recente passaggio da una legge di impianto maggioritario a una prevalentemente proporzionale. Quante volte, per entrare nel merito, cari colleghi, abbiamo detto che, anche mutuando l'esperienza europea, il lavoro del Senato avrebbe tratto giovamento dalla valorizzazione del lavoro in Commissione. Un lavoro svolto lontano dalle tentazioni di un dibattito sotto la luce dei riflettori televisivi, falsato talora dalla comprensibile necessità di parlare più all'esterno di quest'Aula che tra di noi, per un lavoro di stesura legislativo più proficuo possibile. Per questo, la previsione dell'articolo 2, che introduce il criterio dell'assegnazione dei disegni di legge di norma in sede deliberante e redigente rappresenta davvero il migliore contributo in un confronto franco, di merito, ma finalizzato sempre di più a una tempestiva approvazione delle norme e allo snellimento del lavoro parlamentare. Da questo punto di vista, come richiamavano alcuni colleghi, anche la previsione di settimane di lavoro parlamentare interamente dedicate all'approfondimento e alle votazioni in Commissione non solo si riallinea alle migliori prassi europee, ma va incontro alle necessità, che anche tra noi colleghi abbiamo più volte espresso, di un tempo congruo nella sede di approfondimento più naturale, che è la Commissione di merito. In relazione alla riorganizzazione delle Commissioni permanenti, infine, lasciatemi citare l'equiparazione della 14a Commissione politiche dell'Unione europea a tutte le altre Commissioni permanenti e di salutarla come un fatto assolutamente positivo. Chi parla, infatti, è stato promotore, in sede di riforma costituzionale, di norme che valorizzassero, in particolare questo ramo del Parlamento, del Parlamento, quel ruolo di protagonismo rispetto agli atti legislativi dell'Unione europea, nella sua fase ascendente e discendente, che il Trattato di Lisbona affida, in via innovativa, ai Parlamenti nazionali. Per questo, considero la migliore messa a fuoco del lavoro della 14a Commissione come un sostanziale contributo alla specializzazione e alla ulteriore qualificazione di questa Camera. Chi, poi, come il sottoscritto, ha avuto il compito in questi anni di seguire molto da vicino gli aspetti più tecnici del lavoro della nostra Aula non può che dirsi particolarmente soddisfatto delle disposizioni che, nell'articolo 3, vanno nella direzione di semplificare e razionalizzare i lavori del Senato. L'introduzione di sedute uniche, la generale riduzione a dieci minuti dei tempi di intervento dei singoli senatori, la cancellazione dei riferimenti al CNEL, il superamento del voto di astensione come voto contrario e la richiesta del numero legale a inizio seduta, che ormai era diventata mera pratica ostruzionistica, la votazione generalizzata con procedimento elettronico, la nuova disciplina del *question time*, sono tutte scelte che non potranno che migliorare la speditezza e la qualità del lavoro di Aula, favorendo un più proficuo confronto fra maggioranza e opposizione. Vorrei infine richiamare le innovazioni che ricordano anch'esse il dibattito svolto negli anni scorsi sulla Costituzione e su alcuni aspetti della riforma che mi sembra in molti abbiamo condiviso. Mi riferisco in particolare alla possibilità di garantire una corsia preferenziale ad alcune tipologie di atti, in particolare se presentati da minoranze qualificate, che vengono così garantite rispetto alla possibilità di vedere discusse le proprie proposte. In particolare vorrei però citare un istituto di democrazia diretta che in qualche modo già provammo ad inserire nella riforma sottoposta a *referendum* lo scorso 4 dicembre. Grazie al nuovo Regolamento, l'esame dei disegni di legge d'iniziativa popolare dovrà essere concluso entro tre mesi dall'assegnazione e qualora questo tempo passasse inutilmente la proposta sarà iscritta d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea sulla base del testo dei proponenti. Infatti, in un tempo in cui tutti noi siamo impegnati a riavvicinare i cittadini alle istituzioni, a favorire nuovi strumenti di partecipazione che rilancino la nostra democrazia rappresentativa e diano un accesso più diretto al processo legislativo, lasciatemi dire che questa scelta condivisa fa bene a tutti e spero sia tra le cose che insieme rivendicheremo, anche per segnalare agli italiani che la politica e il Parlamento sono decisamente migliori di come, non solo una certa vulgata qualunquista, ma anche noi talora siamo tentati di dipingere, magari per una piccola polemica di parte. Care colleghe e cari colleghi, è davvero un bel segnale concludere questa legislatura con un atto condiviso da tutti i partiti di quest'Assemblea. Siamo certi sarà di stimolo anche alla Camera dei deputati, perché - e vogliamo ribadirlo con il nostro voto - se il Parlamento saprà ritrovare ulteriore efficienza e trasparenza, e con esse una nuova autorevolezza, anche il Paese recupererà un motore di democrazia e di cambiamento attorno al quale riunire le migliori energie e passioni degli italiani, per vincere insieme le sfide straordinarie che attendono tutti noi nei prossimi anni.

Signora Presidente, ho chiesto di intervenire su un'emergenza di cui si parla troppo poco, cioè quella dei suicidi in carcere. Nelle carceri si uccidono i detenuti e gli operatori che vi lavorano. C'è stata una sequenza di casi veramente preoccupante nelle ultime settimane: sabato 9 dicembre si è impiccato nel carcere di Terni un marocchino di trentasei anni ristretto in isolamento perché avrebbe aggredito un agente penitenziario; nella notte dello stesso giorno, nel cercare di massima sicurezza di Tolmezzo, un agente penitenziario di cinquantuno anni si è tolto la vita sparandosi con la sua pistola; e questo era un agente penitenziario. Il giorno precedente, venerdì 8 dicembre, si era impiccato nel carcere di Regina Coeli un sessantenne imputato per ricettazione. Giovedì 7 dicembre (il giorno precedente) una transessuale una transessuale di trentadue anni, in isolamento nel carcere di Rimini, ha tentato il suicidio in segno di protesta e ora sarebbe ancora in rianimazione all'ospedale di Rimini. Anche a fine agosto c'è stata una serie di eventi gravi, gravissimi che, pure oggetto di attenzione da parte del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, confermano una emergenza ancora non adeguatamente affrontata e che vorrei segnalare alla Presidenza. Mi spiace che in questo momento non ci sia alcun rappresentante del Governo, ma spero che la Presidenza possa farsi carico di questa preoccupazione. Il 27 agosto a Monza un recluso si è tolto la vita inalando il gas dalla bomboletta data in dotazione per cucinare; sempre il 27 agosto a Saluzzo un detenuto ha tentato il suicidio in carcere ed è morto poco dopo in ospedale, con il risultato che non risulta morto in carcere, ma in realtà si è suicidato e poi è stato trasportato in ospedale. Sempre a fine agosto ci sono stati due morti in un solo giorno: uno nel carcere di Pisa e un altro a Torino, un croato di ventisette anni. Dall'inizio dell'anno ci sarebbero stati 49 suicidi di persone ristrette, anche se ufficialmente ne risultano di meno perché non vengono conteggiati quelli che muoiono in ospedale

Anzi, gli atti gravi, sempre riportati, nel caso specifico, dalle statistiche del sindacato degli agenti penitenziari, sono molto più consistenti: nei primi sei mesi del 2017, 4.310 atti di autolesionismo tra i detenuti; 3.562 colluttazioni; 541 ferimenti. Per il sindacato le carceri sarebbero più sicure se si assumessero agenti di polizia penitenziaria che mancano:

carenza nell'applicazione della normativa da parte dell'amministrazione sanitaria e dell'amministrazione della giustizia costituisce un grave pregiudizio per detenuti e operatori. La tutela della salute della persona reclusa è riconosciuta dall'articolo 27 della Costituzione - non voglio soffermarmi su tutte le norme che danno attuazione a quell'articolo - oltre che dall'articolo 32, ovviamente, che riguarda tutti gli individui, non soltanto quelli in libertà, e dalle norme che successivamente, a partire dal 1999, e poi nel 2008, hanno finalmente affermato che la salute delle persone ristrette deve essere a carico dell'amministrazione sanitaria, esattamente come la salute di tutte le altre persone che vivono in questo Paese. Recentemente la Conferenza Stato-Regioni ha approvato due provvedimenti proposti dal Governo: un piano per la prevenzione delle condotte suicidarie fra gli adulti e un altro piano per la prevenzione delle condotte suicidarie

un'ultima segnalazione, che è veramente triste. Da poche settimane l'amministrazione penitenziaria ha emanato una circolare che non riguarda questi fenomeni, ma che incide sul clima nel quale si vive all'interno del carcere, momento che siccome le condotte idriche sono dei colabrodi, di chiudere l'acqua dalla sera alla mattina in tutte le carceri e di dotare ogni cella di una tanica con dell'acqua, in modo che la dispersione della stessa e i relativi

indicate. C'è bisogno di un intervento specifico su questo punto. Capisco che a fine legislatura sarà difficile, ma non possiamo trascurare questa emergenza perché è un segno di civiltà per tutto il Paese.

La seduta è tolta